in occasione del dibattito sull'autonomia, avevano denunciato il rischio di partenza anticipata su alcune materie. Molti senatori e molte senatrici, soprattutto senatrici, soprattutto di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, si erano alzati in quest'Aula garantendo a tutte le forze politiche che questa cosa non sarebbe mai avvenuta. Il presidente Zaia ha comunicato formalmente che le materie non LEP riguardanti rapporti internazionali con l'Unione europea, commercio con l'estero, professioni, protezione civile, previdenza complementare integrativa, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, organizzazione della giustizia di pace e - pensi un po', signora Presidente anche il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario possono essere immediatamente trasferite alla Regione. Noi pensiamo che ci sia un tradimento intanto dell'assunzione di responsabilità avvenuta da parte dei Gruppi parlamentari che hanno dichiarato a Palazzo Madama e Montecitorio cose che sono state evidentemente disattese. La richiesta che le rivolgiamo, signora Presidente - e per questo stiamo raccordando tutti i Gruppi di opposizione

sia ancora un punto fermo per questo Governo oppure no. Piaccia o meno, anche le materie non LEP incideranno su quel principio; piaccia o anche le materie non LEP inevitabilmente si portano dietro - presidente Pera - personale e inevitabilmente una quota dei fondi nazionali che vengono utilizzati per la perequazione. Lo diciamo perché è evidente

dare un parere positivo alle richieste che sono arrivate dal presidente Zaia e soprattutto, signora Presidente, ci aspettiamo una presa di posizione della presidente Meloni. Aggiungo che nella giornata di oggi, presidente Ronzulli, è accaduta una cosa molto grave in Commissione giustizia. Mentre le colleghe e i colleghi erano in dichiarazione di voto sul cosiddetto disegno di legge GPA (gestazione

e durante le dichiarazioni di voto si è deciso di sospendere i lavori. Questo è molto grave, signora Presidente, perché ancora una volta, quando la maggioranza si ritrova di fronte alla possibilità di andare sotto, modifica le regole del gioco. Ovviamente tutto questo sarà oggetto di un confronto e di una discussione nella Conferenza dei Capigruppo, che è stata già prevista al termine dei lavori dell'Aula, ma pensiamo che sia inaccettabile. l'ennesima volta che accade un fatto che non è accettabile per la nostra convivenza in quest'Aula. Le regole sono regole, signora Presidente. Se si è in dichiarazione di voto, si vota, anche se si va sotto, indipendentemente dal merito di quell'emendamento. Il presidente Romeo poteva benissimo ritirare quell'emendamento, se fosse stato d'accordo con la relatrice o con il Governo. Se non l'ha fatto, evidentemente è perché non è d'accordo e - guarda caso - c'è un'altra divisione nel Governo. Non si può pensare di nascondere ogni volta le divisioni,

Signora Presidente, nell'associarmi ovviamente alla richiesta che formalizzeremo come opposizioni nelle prossime ore di sentire il ministro Giorgetti rispetto alle richieste che il governatore Zaia ha fatto in queste ore, e quindi nel ribadire la gravità della potenziale attuazione parziale della legge sull'autonomia differenziata, non posso però, senza ripetere - perché le condivido - le considerazioni fatte dal presidente Boccia, non segnalare che siamo in una situazione politica che ha bisogno di un chiarimento. Mi verrebbe da dire, infatti, che forse, invece del ministro Giorgetti, dovremmo interrogare il ministro Musumeci, che ha appena dichiarato che è prematura la proposta fatta dal presidente Zaia e capire se tra il ministro Giorgetti e il ministro Musumeci c'è un coordinamento. Quello che è accaduto in Commissione giustizia, che il presidente Boccia ha appena spiegato all'Aula, è figlio di una divisione politica evidente su un tema sensibile come quello della gestazione per altri all'interno della maggioranza. Non è la prima volta che succede: ricordo su un provvedimento recente l'ipotesi di aumentare i membri di una Commissione durante l'analisi di un provvedimento, perché la maggioranza non reggeva su un emendamento del senatore Lotito. Ricordo quello che sta accadendo in Europa col vice presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, che parla di colpo di Stato, al quale evidentemente partecipa l'altro vice presidente del Consiglio dei ministri, Tajani *(Applausi)*, che supporta ciò che sta succedendo in Europa. Ora è chiaro che c'è una maggioranza che sta litigando su tutto, che si tiene assieme soltanto per la gestione del potere, ma credo che non si possa andare avanti in questo modo e che questa non sia una strada che porta lontano.

Grazie, amministrazione penitenziaria che si occupa della giustizia minorile ha segnalato dei dati *record* di detenuti minori nelle nostre carceri minorili. In tutto questo la linea del Governo è incomprensibile perché il ministro Nordio continua a dire che la visione della pena del Governo non è carcerocentrica ma, è tesa alla rieducazione del condannato, e non parliamo soltanto di sanzioni penali nel senso della carcerazione. però, stiamo parlando di un nuovo reato universale nella Commissione giustizia e ciò che è grave - ed è la ragione per la quale il ministro Nordio deve venire in Senato - è che il Governo oggi sia stato sconfessato

non ha voluto ritirare. Il Governo non è andato sotto, nonostante il relatore e il Vice Ministro abbiano riconfermato che il parere era contrario, soltanto perché, nonostante si fosse in dichiarazione di voto, si è deciso l'accantonamento di un emendamento che si stava votando. Al di là degli aspetti regolamentari molto discutibili, quindi, c'è una questione politica che credo debba essere portata all'attenzione ed essere

del vice presidente Tajani che vota per la Von der Leyen o quella del vice presidente Salvini che fa gruppo con Orban. Insomma, non si capisce più niente. Dato, allora, che la maggioranza di fatto in questo momento non esiste più, perché le linee politiche sono assolutamente contrastanti pubblicamente e oggi - questo è il dato nuovo - anche nelle aule parlamentari, chiediamo che la Presidente del Consiglio venga a spiegarci se è ancora una maggioranza e che il ministro Nordio venga a spiegarci qual è la politica criminale del Governo, perché quello che vediamo con gli atti concludenti è il contrario di quello che lui continua a dichiarare in pubblico.

non si aspetta di definire - come abbiamo scritto - i livelli essenziali di prestazione, che è una cosa - come sappiamo tutti - molto complessa e che a costo zero non è possibile fare; scatta invece il meccanismo per

prima quelle regionali, poi quelle morfologiche, in base a come è conformato il nostro Paese, mettendo in discussione addirittura diritti contrattuali nazionali e non solo e liberalizzando una serie di

l'interrogazione che veniva annunciata. È necessario riaprire questa discussione in modo serio e dire ai cittadini che cosa volete davvero. Non si può, da una parte, sostenere una cosa e, dall'altra, comportarsi in modo davvero

guardata, studiata e letta bene, oppure si è in malafede. Era scritto anche nella relazione del provvedimento che naturalmente la concessione di maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario è subordinata alla

commercio con l'estero, professioni, coordinamento della finanza pubblica e dei tributi, casse rurali, organizzazione dei giudici di pace), non c'era bisogno di ridefinire i livelli essenziali delle prestazioni perché venivano già assodati come garanzia

con delle preintese fatte con l'allora vice ministro Bressa, senza la presenza di una legge quadro che calcolasse i livelli essenziali delle prestazioni, sulle seguenti materie: tutela e sicurezza del lavoro, internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione, commercio con l'estero, territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture, governo del territorio, protezione civile, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, competenze complementari e accessorie, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Sinceramente non riesco a capire, o quantomeno mi dovete far non sono un grandissimo esperto, sono in Parlamento da pochi anni - cosa è cambiato rispetto al 2017 *(Applausi)*, quando, in assenza di una legge che coinvolgeva il Parlamento, il presidente Bonaccini già faceva delle preintese che andavano in questa direzione. Collega Boccia, bisognerebbe riuscire anche a capire cosa c'è di diverso rispetto alla proposta che lei ha fatto quando era Ministro rispetto a una bozza

posso dire io qual è forse la verità, mi sembra di capire da questi movimenti che per la sinistra l'autonomia è buona quando è al Governo e diventa cattiva quando è all'opposizione.

l'Italia. Noi avremo anche i nostri problemini di maggioranza e sensibilità diverse, ad esempio sul tema della maternità surrogata - e a tal proposito invito il Governo a fare una riformulazione che tenga conto della nostra proposta - o sul tema dell'Ucraina. Collega Scalfarotto, noi votiamo per il sostegno all'Ucraina perché siamo siamo convinti, ma chiediamo che accanto - come ho già spiegato bene - ci sia anche un tavolo di diplomazia. Magari, adesso che la pace la vuole anche Zelensky, vi accodate anche voi al treno della pace e della diplomazia, perché sono sicuro che in Italia, per la nostra storia, succede sempre così. Avremo anche i nostri problemini e sensibilità diverse all'interno della maggioranza, però, se posso dirvelo, voi dell'opposizione siete semplicemente ridicoli.

la finalità di questo provvedimento è quella di consentire concretamente il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari. Disciplina altresì la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza. Viene puntualmente regolata la materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per queste associazioni. Sono apportate modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Viene incrementato il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa. Si vuole premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate, nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata la difesa. Infine, il provvedimento in esame comprende una disposizione volta a garantire la copertura finanziaria necessaria al finanziamento del NATO Innovation Fund per l'anno 2024. Questo decreto-legge si inserisce all'interno del perimetro tracciato dalla legge del 28 aprile 20233, n. 46, legge che ha definito l'ambito nel quale è possibile istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Voglio ricordare che è del 2018 la sentenza della Corte costituzionale n.120 che va a modificare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di diritti sindacali dei militari. Per la prima volta veniva riconosciuta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale. Era il luglio del 2023 quando, come Gruppo Fratelli d'Italia, interrogammo il Ministro della difesa, l'onorevole Crosetto, su quali azioni il Governo Meloni intendesse muoversi in questo ambito. Sono soddisfatta di aver potuto allora interrogare il Ministro personalmente e oggi di essere relatore di questo provvedimento.

Signor Presidente, il provvedimento in questione ha come fine quello di poter consentire al personale militare il pieno svolgimento delle attività sindacali e questo in piena attuazione di un diritto peraltro riconosciuto anche con una sentenza della Corte costituzionale. Regolare e quindi riconoscere la legittimità dell'esercizio dei diritti sindacali in ambito militare e, al contempo, tutelare l'operatività delle Forze armate era evidentemente una priorità per creare tutte quelle condizioni per i nostri uomini e le nostre donne in divisa per operare al meglio all'interno di un quadro normativo di sicurezza per la salvaguardia dei loro diritti. È un passaggio essenziale, in particolar modo in un momento dove le Forze armate ricoprono un ruolo sempre più importante e strategico, in un contesto globale caratterizzato da instabilità e incertezza. Il ruolo dei nostri militari sarà sempre più importante ed è quindi necessario che la politica ascolti attentamente le loro richieste per capire dove e come poter intervenire per garantirne la massima operatività. In questo senso va sicuramente un'altra importante disposizione, citata anche dal relatore, del provvedimento in esame: quella descritta all'articolo 4, in cui si incrementa di ulteriori 6.650.000 euro il fondo della spesa, che ammonta già a un milione, autorizzata dalla legge di bilancio 2004, al fine di far fronte agli impegni derivati dalla sottoscrizione del NATO Innovation Fund. In un'epoca in cui dobbiamo affrontare non solo le minacce tradizionali ma anche quelle ibride provenienti da domini come quello *cyber* e dallo spazio, è necessario sostenere chi fa innovazione nel campo della Difesa e dare a quelle imprese, anche piccole e medie o *startup*, la possibilità di operare all'interno del quadro delle alleanze tradizionali e atlantiche, onde soprattutto evitare di avere dei Paesi *competitor* o addirittura ostili, più all'avanguardia di noi in settori strategici e tecnologici. Inoltre, non non bisogna assolutamente sottovalutare l'impatto duale di queste tecnologie, che possono avere ricadute anche sulla vita civile oltre che su quella militare.

compiendo quindi significativi passi in avanti per garantire i diritti sindacali in ambito militare.

2022, che dispone le norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate. Questo - come è stato peraltro ricordato dalla relatrice nasce a seguito di un'importante sentenza della Corte costituzionale, la n. 120 del 2018, che stabilì di fatto, invertendo un principio tradizionale assodato, che era possibile costituire all'interno delle Forze armate associazioni professionali a carattere sindacale. Tutto questo avviene all'interno di un quadro che muta, tra l'altro, in circostanze particolari. In questo decreto non c'è soltanto la vicenda delle associazioni professionali professionali a carattere sindacale all'interno delle Forze armate, ma vi è anche - lo ricordava poco fa il collega Dreosto - una norma importante dedicata al al sostegno delle *startup*, cioè investimenti in termini di sviluppo e tecnologie emergenti che riguarda la partecipazione dell'Italia al Fondo multisovrano di *venture capital*, che è denominato NATO Innovation Fund, per

i venti di guerra spirano su più fronti; in cui vi sono vicende di carattere internazionale e in cui si ridisegna lo scacchiere a livello tanto globale quanto regionale, e dunque spesso il fatto di esserci, di essere comunque presenti. Questo è un altro dei temi assolutamente all'ordine del giorno. Sulla prima questione noi riflettiamo intorno al fatto che è cambiato un quadro che storicamente era fissato.

di una presenza sindacale all'interno del mondo militare. Cioè quanto era ed è compatibile per davvero che

inserita all'interno del dettato costituzionale come sacro dovere del cittadino di difendere la Patria. Su tante cose si riflette ultimamente

Penso che non sarebbe così folle se ci si ricominciasse a interrogare sulla sua opportunità anche per il nostro Paese, come stanno facendo Paesi *partner* europei, tanto in ambito

2024 per la quantificazione del contingente dei distacchi e permessi prevista dalla contrattazione. Questo perché si tratta per il momento, almeno in questa indicazione numerica e tecnica, di una norma che va considerata fino al

nel precedente esercizio di bilancio dello scorso anno si era previsto un intervento italiano di otto milioni; attualmente abbiamo impegnato solamente un milione nonostante l'impegno italiano fosse di 7.650.000 per anno. articolo quindi non fa null'altro che rendere il nostro impegno in termini di bilancio effettivo per ciò che riguarda il contributo italiano. Si tratta quindi di un decreto-legge che ha oggettivamente carattere di urgenza per intervenire soprattutto in queste due particolari questioni, sulle quali ovviamente non possiamo che che trovarci d'accordo con la formulazione originaria del Governo e anche con gli interventi parziali che sono passati attraverso il primo ramo del Parlamento.

di ricordare che sono trascorsi trentuno anni dalla tragica battaglia del *checkpoint* Pasta a Mogadiscio. Il 2 luglio 1993 miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto l'egida ONU, per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione somala, costretta alla fame e alla sofferenza per le lotte fra le fazioni tribali. Tre giovani e valorosi militari italiani, il sottotenente Andrea Millevoi,

il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare, *(Applausi)*, che, nonostante abbia riportato gravi infortuni da quel terribile attentato, ancora oggi con la sua passione e la sua dedizione concorre alle attività volte a sostenere il Dicastero della difesa. Questo provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano materie di importanza e di interesse per il Ministero della difesa. In particolare, rispetto alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari (ovvero i sindacati), permette, con il finanziamento del contingente di distacchi e permessi, di poter svolgere quell'attività di contrattazione che in questo momento è in corso. Ricordo che il Governo ha stanziato per il comparto difesa e sicurezza un miliardo e 400 milioni per il rinnovo del contratto del triennio 2022-2024 per cui era necessario finanziare anche i distacchi e i permessi in modo che le sigle sindacali potessero esercitare le proprie funzioni. Allo stesso tempo, era anche importante allineare le soglie di rappresentatività con le Forze di polizia ad ordinamento civile.

13.000, fra donne e uomini, che svolgono un lavoro straordinario a servizio del Dicastero cui va, insieme alle nostre Forze armate, un profondo senso di gratitudine e di ringraziamento. Un altro aspetto importante di questo provvedimento, proprio perché viviamo in un contesto di conflitto ibrido di importanza delle nuove tecnologie, soprattutto nei settori della *cybersecurity* e dello spazio, è il finanziamento di ulteriori 6 milioni di euro per il NATO Innovation Fund, un fondo di *venture capital*, il più importante importante fondo costituito a sostegno delle *startup*. Per un Paese come il nostro, il cui tessuto economico è per lo più caratterizzato da piccole e medie imprese, è importante finanziare questo fondo. L'impegno del Governo, complessivamente distribuito negli anni, è di 80 milioni di euro, proprio perché

ai settori dello spazio e della *cybersecurity*). Complessivamente si tratta di un provvedimento che va a redigere alcune norme che sono fondamentali per l'esercizio delle funzioni. Ricordo, in conclusione, che si è passati dalla rappresentanza ai sindacati; questo è frutto anche dell'approvazione della legge n. 46 del 2022, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale. Per cui ci troviamo in un nuovo regime, quello dei sindacati, a cui

contemporaneamente, nel maggio 2024 il Governo ha fatto un decreto che ha disciplinato, con una normativa di uguale rango, la stessa identica cosa, creando di fatto una confusione interpretativa. Quale delle due è vigente? Con l'emendamento 1.0.2 abbiamo previsto la scadenza nell'articolo della legge di bilancio, al pari di quello che prevede il decreto. Ciò per evitare qualsiasi dubbio. È vero che gli effetti del comma della legge di bilancio scaduti il 30 giugno (quindi due giorni fa), ma è possibile che tutte le volte il Governo non preveda la disciplina dell'abrogazione esplicita e lasci contemporaneamente vigenti

idonee risorse per rendere strutturale l'incremento del Fondo anche per le successive annualità.

Istituzionalmente è un ordine del giorno che viene approvato. l'ordine del giorno può essere accolto. L'impegno del Governo rispetto alla materia c'è stato quest'anno. Infatti, stiamo parlando di un decreto che finanzia 10 milioni di euro sul fondo risorse decentrate per personale civile della difesa.

questo è un fondo che ha creato il Governo Conte, quindi in teoria siamo anche favorevoli. Il discorso è che non c'entra assolutamente nulla con questo decreto-legge. Anche qui c'è il malvezzo di continuare a inserire

Signor Presidente, questo provvedimento costituisce un passo in avanti decisivo rispetto a un percorso che è iniziato nel 2018 con una sentenza della Corte costituzionale, che ha finalmente dichiarato illegittimo il divieto delle Forze armate di organizzarsi in associazioni sindacali. Il percorso è poi proseguito nel 2022 con la legge quadro, fino ad arrivare a questo provvedimento. provvedimento. È importante spiegare ai nostri concittadini il significato profondo di questo nostro provvedimento, volto a strutturare e potenziare la rappresentanza sindacale delle Forze armate. Innanzitutto è una questione di buon senso: i militari sono lavoratori e meritano, come ogni lavoratore, ampie garanzie di assistenza e una piena valorizzazione del loro operato. In altre parole, tutti i santi giorni le Forze armate mettono in gioco non solo la propria esperienza e professionalità, ma anche la propria vita per difendere la nostra sicurezza rendere l'Italia un Paese migliore. Quindi, il minimo che si possa fare è impegnarci a nostra volta a difendere la loro sicurezza sul lavoro, migliorando le premesse alla base della loro attività, troppo spesso bistrattata e misconosciuta. Equiparare la rappresentanza sindacale delle Forze armate in Italia agli *standard* europei e migliorare la sicurezza e la trasparenza sono due obiettivi che questo provvedimento si prefigge di ottenere, così come l'importanza di un principio di imparzialità delle sigle sindacali delle Forze armate, in linea con quanto è stato sancito dalla legge del 2022. Quindi, direi che questo è un provvedimento doveroso che va nella giusta direzione e che all'articolo 1 prova a garantire una prerogativa costituzionale, quella dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti anche per i rappresentanti delle associazioni professionali delle Forze armate; all'articolo 2 prevede invece un adeguamento del processo di revisione della rappresentatività a livello nazionale dei sindacati delle Forze armate. Quello che è ancora più importante è che all'articolo 3 viene stanziata una cifra

per il 2024 in favore del NATO Innovation Fund, un fondo di *venture capital* per l'innovazione nel settore della Difesa e di cui l'Italia è il terzo investitore investitore ed è proprio il NATO Innovation Fund che ci aiuta ad arrivare al nocciolo della questione: investire in questo fondo significa investire in *startup*, in tecnologie

più bisogno oggi, in un frangente storico così incerto e travagliato. Per tutte queste ragioni, noi di Azione voteremo a favore del provvedimento. Si tratta di un voto improntato ad una logica di buonsenso, di responsabilità e di interesse comune. Prima di concludere, voglio ringraziare tutti i rappresentanti delle Forze armate per il lavoro benemerito che svolgono e per i tanti, troppi rischi che corrono ogni giorno al fine di aiutare, difendere e proteggere i cittadini del nostro Paese. Alle donne e agli uomini in divisa dobbiamo la tutela della nostra sicurezza, che è presupposto della democrazia in cui viviamo e della libertà di cui anche per merito loro godiamo tutti incondizionatamente.

ci sono donne e uomini che antepongono ai propri interessi quelli degli altri, donne e uomini che indossano una divisa e sono pronti a sacrificare la propria vita, donne e uomini che tutelano gli altri prima che sé stessi. Eppure, nella nostra Italia a loro fino ad oggi non era riconosciuto un diritto costituzionalmente garantito. Parliamo di diritti che, soprattutto a chi tiene alto il nostro Tricolore in Patria e all'estero, riguardano l'associazionismo sindacale, uno strumento di autotutela e di benessere lavorativo e professionale che proprio nel personale militare dovrebbe essere assicurato pienamente. Oggi in quest'Aula, dopo l'approvazione alla Camera, finalmente possiamo mettere fine a un *vulnus* incomprensibile. Con questo provvedimento, presentato dal presidente del Consiglio Meloni e dal ministro della difesa Crosetto, siamo qui chiamati al nostro dovere di garantire a tutti gli italiani, a prescindere dalla professione, i medesimi diritti. n. 61 del 2024, infatti, reca disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. Anche per loro, con l'auspicio che tutta l'Assemblea di Palazzo Madama, con ogni forza politica, al di là del proprio orientamento, dia il proprio sostegno a questa importante misura, sarà prevista la possibilità di avere strumenti di autotutela ricorrente all'associazionismo sindacale. 46 del 28 aprile 2022 ha rappresentato un primo passo in questo senso, ma era pur sempre solo destinata a delineare un quadro più ampio. Con il decreto che oggi ci accingiamo a convertire di riconoscere dei diritti ai nostri militari, in linea con gli *standard* dell'Europa. Si tratta di un riconoscimento dovuto a coloro i quali, nonostante l'impegno, la passione, la dedizione, l'onore, questo diritto non era concesso, ma che anzi si ritrovavano a essere vittime di attacchi verso un ruolo troppo spesso sminuito, dimenticato, criticato e contrastato. Questo è un traguardo a cui lavoriamo da tempo ed era inevitabile e doveroso dare piena attuazione della legge n. 46 del 2022, che ho prima citato, attraverso un provvedimento specifico voluto fortemente dal Governo Meloni, un Esecutivo che ascolta e dà risposte concrete senza falsi e vuoti annunci, dimostrando la volontà di sostenere un comparto fondamentale per la sicurezza delle nostre vite e che si pone come un presidio imprescindibile in difesa della nostra democrazia. Non si tratta solo di sindacati che opereranno per promuovere in senso classico la salute dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma forniranno assistenza fiscale e attività di consulenza, disciplinando e regolamentando, ad esempio, tra le altre, la materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti, assicurando inoltre quegli strumenti necessari per svolgere il proprio mandato con efficacia. Saranno infatti incrementati gli stanziamenti per il fondo risorse decentrate per premiare la produttività di chi, con impegno quotidiano e dedizione, garantisce il funzionamento delle Forze armate. Non potevamo continuare a far finta di niente, come se non ci fosse una tale non ci fosse una tale zona d'ombra proprio nei confronti di chi, con elevatissima professionalità, coraggio e fermezza, rappresenta un'eccellenza della nostra Nazione. Lavorare per rafforzare i diritti di tutti è un dovere e un obbligo morale. È quindi bene concentrarsi su investimenti per il settore, puntando su tecnologie e sviluppo, ma per avere Forze armate all'altezza, c'è la necessità di garantire a questi lavoratori tutti diritti, senza alcuna pregiudiziale priva di fondamento. Il nostro ringraziamento a coloro che quotidianamente ci difendono passa anche attraverso l'approvazione del provvedimento

brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. Come è stato ampiamente ricordato, la sua finalità principale è dare concreta attuazione a un diritto, quello all'attività sindacale, riconosciuto da una sentenza della Corte e da un successivo intervento legislativo della scorsa legislatura. Con il provvedimento in esame si compie il passo successivo, integrando il piano normativo con disposizioni volte al fattivo esercizio di questo diritto; penso, quindi, al diritto ai distacchi e ai permessi retribuiti, senza i quali nessun rappresentante sindacale potrebbe svolgere efficacemente la propria attività. è poi la modifica alla normativa sulla rappresentatività delle associazioni sindacali, che abbassa la percentuale degli iscritti richiesti, per venire incontro al fatto che ad oggi solo il 15 per cento delle forze militari ha aderito alle rappresentanze sindacali. Su questo, come si è detto in Commissione, serve un intenso lavoro per garantire lo sviluppo di un sano pluralismo: più soggetti sindacali ci sono, naturalmente fondati su una base concreta di iscritti, migliore è la rappresentanza degli interessi e dei bisogni dell'intera categoria.

dovrà servire soprattutto a sviluppare quei progetti legati a una condizione difensiva e possibilmente non offensiva. In conclusione, signora Presidente, il provvedimento in perché guarda ai militari nel loro essere lavoratrici e lavoratori di un settore chiave dell'interesse nazionale. Colgo quindi anch'io l'occasione per ringraziarli e per esprimere gratitudine verso quelle persone in divisa impegnate in missioni all'estero e per tutti quelli che, con la loro professionalità e il loro impegno, ogni giorno tengono alti i nostri valori, a cominciare da quello della pace. Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie sul provvedimento in discussione. la mia dichiarazione di voto, sul merito, sarà molto breve. Questo è un voto favorevole, da parte del mio Gruppo. Tutte le norme che vanno a sostenere le attività delle nostre Forze Armate meritano di essere guardate con grande attenzione. I colleghi che mi hanno preceduto hanno sottolineato l'importanza, anche il ruolo fondamentale, nella vita democratica del Paese, il prestigio internazionale che le nostre Forze Armate hanno nel mondo. Quindi, non c'è motivo di votare contro. Però, chiedo ai

di permessi e di rappresentatività delle sigle sindacali. Ricordo che chi le parla ha un passato di direttore del personale. Questo atto poteva star bene dentro una circolare ministeriale o poco più. Io mi chiedo davvero come si possa pensare che gli articoli 76 e 77 della Costituzione consentano al Governo di riunirsi e di emanare un provvedimento avente immediatamente forza di legge su una materia così regolamentare. Ci sono poi anche delle questioni finanziarie, che rispetto. Però, la funzione legislativa del Parlamento è sottratta a queste Camere per certe Io cerco anche di fare il mestiere dell'opposizione, cercando qualcosa da criticare. Ma che cosa devo criticare, se si parla della rappresentatività delle sigle sindacali delle Forze armate? Come appunto diceva il collega Spagnolli, sono dei lavoratori e delle lavoratrici ed hanno diritto, come ha detto la Corte costituzionale, di svolgere attività sindacale. Però, io ricordo sentenze della Corte costituzionale che danno delle indicazioni cui il Parlamento non ha dato seguito. Si pensi a tutto il fine vita; pensi a tutto il tema dei figli delle coppie omosessuali. La Corte costituzionale, come il presidente Barbera ha ricordato da poco, ci dice che dobbiamo legiferare e noi non legiferiamo. Invece, il Governo che cosa fa? Si riunisce per adottare un provvedimento di straordinaria necessità

Mi viene da chiederle, signor Sottosegretario, ma per quale motivo non avete fatto presentare alla collega Zedda (anzi, al collega Zedda, non vorrei mai sbagliare l'identità di genere del collega)

*ex* articolo 77 così ordinamentali, in realtà è un'umiliazione che diamo alle istituzioni. Una umiliazione che, in questo caso, è proprio gratuita, non serve a niente, non aggiunge niente a voi e toglie alle Aule di questi Palazzi così importanti, che rappresentano più di quello che pensiamo.

alle decisioni che prende il Governo. Questo è il dato fondamentale. Questa è la ragione per la quale, proprio su questo punto dovrei dire che siamo contrari. Per questa ragione ci asterremo dalla dalla votazione, perché nel merito nessuno di noi mette in discussione la necessità di dare un'organizzazione sindacale ai militari, però questo è il dato di fatto.

che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. Noi siamo contrari a questa cosa e siamo molto perplessi sull'utilizzo di questo Fondo. Per questa ragione abbiamo

ovviamente con regole discendenti e attagliate alle peculiari e delicatissime attività svolte dalle Forze armate nell'interesse dello Stato e allo stesso tempo dei cittadini. Ci sono voluti molti anni per arrivare alla costituzione delle associazioni sindacali militari. Tengo a ricordare che nel 2018 c'è stato un pronunciato innovativo della Corte costituzionale che ha aperto la strada a una disciplina puntuale per regolamentare la complessa e inedita tematica dell'associazionismo sindacale tra militari, che è forse diversa e peculiare da quella che riguarda altri lavoratori, proprio per lo specifico *status* giuridico degli uomini e delle donne in uniforme del Ministero della difesa. Al termine della precedente legislatura la legge n. 46 del 2022, a lungo esaminata e discussa, per la prima volta ha stabilito in Italia norme per regolare esercizio della libertà sindacale del personale militare. Le regole riguardano quindi l'associazione tra militari che deve essere libera, volontaria e individuale. Le associazioni di questo tipo devono vivere nella massima trasparenza dei contributi sindacali degli iscritti e delle attività della gestione, che prevede anche la consulenza e assistenza fiscale a favore degli iscritti. Si è quindi reso necessario un decreto-legge per adottare disposizioni che assicurassero il pieno esercizio delle attività professionali di carattere sindacale, ma anche per garantire una maggiore funzionalità del personale militare del Ministero della difesa, così come la massima operatività delle Forze armate. In particolare, sono adesso definite anche le modalità di partecipazione alle associazioni professionali a carattere sindacale e alle procedure di contrattazione del comparto difesa e sicurezza. Inoltre sono regolamentati in modo attento i distacchi e i permessi sindacali retribuiti. Viene altresì puntualizzata quella che è una disciplina transitoria che riguarda la rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale militare. L'idea è che, trattandosi di associazioni in via di costituzione, vi debba essere una progressività per raggiungere il livello di rappresentatività,

A tal proposito si è pensato ad un meccanismo di progressività simile a quello che è stato già adottato in anni passati quando furono costituiti i sindacati della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria. Nel provvedimento in questione ci sono anche disposizioni che riguardano più prettamente l'operatività della Difesa. Viene infatti incrementato il fondo risorse decentrato dal personale civile di ulteriori 10 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio. Vale ricordare che la delega di revisione dello strumento militare aveva previsto la razionalizzazione della dotazione organica civile della Difesa a 20.000 unità entro la fine di quest'anno, dalle quasi 28.000 in essere nel 2012. È presente poi l'aumento del finanziamento del fondo di *venture capital* NATO Innovation Fund, destinato a sostenere l'avvio di imprese che sviluppano soluzioni tecnologiche all'avanguardia in termini di difesa e sicurezza. I senatori di Forza Italia voteranno guardando con favore al provvedimento che ancora una volta mira alla riorganizzazione di un comparto fondamentale della vita democratica dell'Italia; un provvedimento che punta alla soddisfazione degli interessi di chi mette la propria competenza a disposizione di un lavoro difficile a difesa dello Stato e al quale si chiede di andare incontro a nuove sfide. avviene in un contesto in cui si ragiona di difesa europea, che comporta un modello organizzativo più collegato tra gli Stati europei con le economie di scala e gli efficientamenti organizzativi e logistici che questo porta con sé all'interno dell'Alleanza atlantica. Si tratta di un modello che immaginiamo

anzitutto attuando e modificando una legge fortemente voluta e scritta dal MoVimento 5 Stelle. È il segno che il MoVimento 5 Stelle ha caratterizzato gli ultimi anni della politica italiana con riguardo alle associazioni sindacali per i militari, fortemente volute dopo la sentenza della Corte costituzionale. In quel periodo io non ero parlamentare, ero in forza al Governo e ricordo che è stato un compito estremamente difficile. Avrei fatto scelte anche differenti, ma credo sia stato il compromesso migliore possibile con gli strumenti dati in quel periodo. Quindi, siamo molto orgogliosi di quello che è stato ottenuto.

soprattutto in virtù del fatto che questo provvedimento poteva essere fatto con un altro strumento normativo, come già ampiamente descritto dal senatore Scalfarotto. Io mi domando - come ho già detto prima in dichiarazione di voto sull'emendamento - di quale schizofrenia sia ormai preda il Governo, che vuole legiferare con decreti d'urgenza su qualsiasi cosa. Credo che sia il momento di fermarsi e di iniziare di iniziare a ragionare in termini diversi, coinvolgendo il Parlamento o comunque i Ministeri, quando di competenza. In secondo un aspetto positivo è stato l'accoglimento dell'ordine del giorno che aumenta i fondi per il personale civile. Ma faccio presente che in audizione le parti sociali del personale civile del comparto comparto Difesa hanno evidenziato la situazione drammatica del personale, che era previsto in diminuzione a 20.000 unità, ma che già oggi conta 11.000 unità se ben ricordo - comprendendo i 3.000-4.000 che sono transitati dal personale militare a quello civile. Siamo di fronte a una carenza di personale enorme. enorme. Mi domando allora: se, invece di spendere tutti i soldi che abbiamo speso in armamenti e in nuovi programmi di armamento, si pensasse prima al personale, non si farebbe una cosa migliore? Non sarebbe cosa migliore migliore attuare un miglioramento del personale? Pongo qui la stessa domanda che ho posto al ministro Crosetto in audizione l'anno scorso: come pensate di rendere appetibile il reclutamento al Ministero della difesa di personale altamente qualificato in termini *cyber*, ad esempio, quando, con le norme vigenti, ci sono tetti di spesa per il personale e inquadramenti ben precisi, che le aziende private non hanno, che possono tranquillamente competere con il Ministero, portandosi a casa le migliori menti? Credo che questa sia una riflessione da fare. Probabilmente è giunto il momento di cambiare anche la legge sul reclutamento del personale militare militare e civile. Abbiamo bisogno di professionalità elevate. Credo che sia il momento di cambiare le regole, affinché sia appetibile essere reclutati al Ministero della difesa.

rappresentatività delle forze sindacali. Ora, è notizia che dovrebbero sapere tutti - e immagino la sappia anche il Sottosegretario - che la settimana prossima, il 9 luglio, il TAR del Lazio dovrà esprimersi

perché non è stata applicata la stessa rappresentatività che viene applicata alle Forze di polizia. È stato previsto nella legge - e questo è uno degli errori di cui parlavo prima - che la rappresentatività sia calcolata sulla forza effettiva in essere, mentre nelle Forze di polizia è calcolata

ha ragione il sindacato: non è possibile, allo stato attuale, definire rappresentativo al 2, al 3 o al 4 per cento - scegliete voi la proporzione di tutta l'intera forza del personale, quando la parte sindacalizzata non arriva credo al 10 per cento del totale. Credo che ci sia ancora il timore di aderire alle organizzazioni sindacali, perché evidentemente il Ministero della difesa, la gerarchia che vige nel Ministero della difesa incute ancora timore nell'esporsi e candidarsi a ruoli

questi casi: sarebbe il caso di adeguarsi alla stessa normativa che vale per le Forze di polizia, visto che avete scelto lo stesso lasso temporale per arrivare alla contrattazione, sacrosanta, al 31 dicembre 2024, e di applicare quanto meno le stesse regole. Signor Sottosegretario, credo che si poteva fare molto meglio e con strumenti differenti. Noi, come MoVimento 5 Stelle, eravamo disponibili quando abbiamo scritto la legge; siamo disponibili a migliorarla e siamo disponibili tutt'oggi a cercare di porre un rimedio a quanto detto prima per il personale e a sistemare anche le incongruenze che state reintroducendo con il decreto-legge in esame. Pertanto, annuncio nuovamente l'astensione, nella speranza di poterci sedere a dei tavoli

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il punto cruciale della riforma che tra poco andremo ad approvare è quello di garantire l'esercizio dei diritti sindacali in ambito militare e, al tempo stesso, tutelare l'operatività delle Forze armate. Si tratta di complesso che ha visto un lungo percorso nella scorsa legislatura per la nascita di una legge sui sindacati militari. L'esigenza di legiferare su questo tema nasce a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2018, del 2018, che ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, dove si stabilisce il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, con la necessità quindi che le associazioni siano composte solo da militari e che le stesse non possano aderire ad associazioni differenti. La sentenza ha stabilito, tuttavia, la legittimità riguardo al divieto per i militari di scioperare, precisamente al comma 4 dell'articolo 1475 del codice di ordinamento militare. La sentenza della Corte costituzionale ha ribadito tuttavia come ho già riferito - alcune norme che delimitano un perimetro e ha di fatto delegato il Parlamento a stabilire i tempi e le modalità per regolamentare la nuova disciplina. L'*iter* ha visto la sua conclusione con l'approvazione della legge n. 46 dell'aprile 2022, al cui esito hanno lavorato tutti i Gruppi parlamentari attraverso molteplici audizioni e una mediazione necessaria fra le parti. La legge prevede una delega al Governo per il coordinamento normativo, fornendo il quadro giuridico in cui è possibile istituire per la prima volta nell'ordinamento italiano associazioni professionali a carattere sindacale fra i militari. Oggi quindi con il voto al decreto-legge in esame consentiremo il primo concreto svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra i militari, disciplinando altresì la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari e le procedure di contrattazione del comparto difesa e sicurezza, regolamentando in modo più circostanziato la materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per queste associazioni. Ringrazio, per suo tramite, Presidente, i Cocer per il lavoro svolto fino ad ora. Da parte di tutto il Gruppo, faccio gli auguri anche alle associazioni neocostituite per il prosieguo dei prossimi lavori congressuali. Un altro elemento contenuto nel decreto-legge che a breve voteremo riguarda l'articolo 3, e precisamente la previsione di 10 milioni da destinare all'incremento del Fondo per le risorse decentrate del personale civile non dirigenziale; incremento deciso a fronte del numero crescente di compiti e funzioni svolte proprio dal personale civile della Difesa che supporta le Forze armate. Anche il personale civile soffre dei tagli stabiliti dalla legge n. 244 del 2012 e li soffre in maniera ancora più accentuata, essendo numericamente insufficiente a far fronte a tutto ciò necessario per garantire il supporto alla capacità operativa delle Forze armate. Ringrazio il Governo per aver accolto mio ordine del giorno, che dà la possibilità di prevedere che il fondo dei 10 milioni che è stato stabilito possa essere reso strutturale. Mi lasci ringraziare, signora Presidente, per suo tramite, tutti gli uomini e le donne delle Forze armate che ogni giorno antepongono la difesa della Patria *(Applausi)* e di tutti noi alla loro stessa vita, con senso di responsabilità e spirito di sacrificio, sacrificio a cui spesso sottopongono le loro famiglie. Grazie quindi a loro, famiglie comprese. famiglie comprese. Prima di chiudere, di fronte alle lezioncine da parte di qualcuno su quelle che sono le cose che avremmo potuto fare maggiormente nei confronti del personale militare e civile come ho sentito nell'intervento che mi ha preceduto del collega Marton - io direi che l'interesse del MoVimento 5 Stelle nei confronti del personale militare e civile l'abbiamo visto in atti concreti. In un momento in cui il Ministro della difesa è stato il loro non ci sono stati atti a supporto è la legge che posticipa di nove anni l'entrata a pieno regime della legge n. 244 del 2022. Quindi, lezioni da chi, nel momento in cui aveva la possibilità di farlo, non ha fatto nulla non le accetto.

importante e dovuto. Abbiamo poi molte perplessità - lo dirò più tardi - sul modo con cui si arriva alla conclusione, ma senz'altro il fatto di dare applicazione alla legge n. 46 del 2022 e, quindi, di recepire in maniera piena l'indicazione della Corte costituzionale, che nel suo pronunciamento ha modificato l'orientamento che aveva avuto sempre, riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale, è una una positiva evoluzione. Ne prendiamo atto: è un'evoluzione che riconosce l'altissima professionalità delle nostre Forze armate, che sono fatte da grandi professionisti e da persone competenti, che difendono l'ordine, la sicurezza e anche un'idea dell'Italia protagonista nelle mediazioni. Penso al Kosovo, penso al Libano; penso alle esperienze in cui i corpi militari italiani si sono contraddistinti per la loro saggezza e la loro capacità di trovare ragioni di dialogo e di convivenza, anche laddove queste sembravano impossibili.

ripeto - noi avremmo voluto contribuire in maniera più importante a questo provvedimento. Noi abbiamo proposto nel nostro emendamento che l'indennità accessoria del personale fosse estesa non solo al personale civile ma anche al personale militare. Purtroppo qui ci sono solo 10 milioni del fondo risorse decentrate per il personale civile e non ci sono per il personale militare. Avevamo chiesto - spero che il

che si debba riunire un Consiglio dei ministri con un Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i Ministri del Governo per fare un decreto su dei distacchi sindacali appare veramente una cosa che non ha né capo né coda. *(Applausi)*. benissimo prima di me il senatore Scalfarotto l'ha detto il senatore Marton; lo ha detto il senatore Magni. Non è un problema dell'opposizione, però, signor Sottosegretario: questo è un problema del Parlamento ed questo è un problema del Parlamento ed è un problema di dignità. Si poteva fare un disegno di legge, discutere, magari anche affrontare altri argomenti collegati a questo, ma non certamente introdurre

Se questo è un decreto che parla di distacchi sindacali, di normative che potevano benissimo essere fatte in maniera differente, comunque si poteva fare un disegno di legge ed evitare un'inutile umiliazione al Parlamento. Mi sto chiedendo perché

comunque i provvedimenti legislativi perderanno sempre di più qualità ed efficacia. È evidente, infatti, che il Governo non può esaurire dentro le sue strutture o per mano dei capi degli uffici legislativi dei Ministeri la capacità e la complessità degli argomenti. argomenti. Continueremo ad avere provvedimenti che devono essere presi così come sono o niente e continueremo ad avere un impoverimento della proposta legislativa del nostro Paese: mi sembrano due elementi innegabili, oltre all'umiliazione ormai palese del ruolo di questa Ho una certa età e quindi potrei anche essere felice di essere pensionato anticipatamente, e cioè di essere considerato uno che si deve riposare. Ma, siccome vengo pagato per lavorare in quest'Aula e possibilmente anche per contribuire al bene del mio Paese, vorrei che il Governo si ricordasse che ci sono centinaia di persone che dovrebbero svolgere il ruolo che oggi il Governo si è arrogato su un argomento assolutamente non pertinente, visto che il Governo stesso avrebbe cose molto più serie di cui occuparsi.

cui risultanze andranno a ricadere su un numero non esiguo di italiani appartenenti alle nostre Forze armate: sono oltre 160.000 del nostro comparto difesa diviso tra Esercito, Aeronautica, Marina; oltre 100.000 carabinieri e 60.000 finanzieri. di un mondo che, tra l'altro, credo sia spesso la parte migliore dell'Italia, e non solo all'interno dei nostri confini nazionali, ma anche e soprattutto all'estero.

il tricolore formalmente sul braccio ma sostanzialmente nel cuore, difendono e rappresentano l'Italia quotidianamente, raccontano l'Italia migliore, quella che proprio grazie alla loro azione sullo scenario internazionale viene apprezzata. Non a caso l'Italia

Tutto questo non serve solo per metterci una cosiddetta medaglia sul petto, ma serve anche per difendere anche e soprattutto l'interesse nazionale all'estero. Allora anche con le nuove missioni, come la missione Levante e la missione Aspides, che dal 2024 si aggiungono alle 40 già in corso nell'anno precedente, queste persone e quelle che quotidianamente o a intervalli regolari si alternano nelle loro missioni meritano e meritavano alcuni riconoscimenti anche da un punto di vista meta-giuslavoristico e sindacale, per poter difendere al meglio le loro condizioni.

svolgere attività assistenziali, culturali, attività di inserimento nel mondo del lavoro per coloro i quali dovessero invece abbandonare la carriera o il mondo militare. Sono sicuramente tutte cose positive che però, giustamente, vengono bilanciate vista la particolarità di un mondo che deve avere delle peculiarità che lo differenziano dalle altre organizzazioni sindacali.

cosiddetto mondo civile. Io credo che questa sia una normativa di buon senso che bilanci gli interessi dei dipendenti, siano essi del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze, delle nostre Forze armate e di alcune peculiarità proprie dell'indossare una divisa che, evidentemente, pone delle priorità diverse rispetto ad altri tipi di dipendenti. Credo che questa normativa raggiunga un bilanciamento di livello complessivamente molto alto e che ciò non era ancora stato fatto in passato. A me fa piacere che una parte dell'opposizione voterà a favore del provvedimento

forse, le tempistiche non sono state le più rallentate della storia del Parlamento italiano, ma nessun dibattito è stato soffocato. Abbiamo analizzato gli articoli. A coloro i quali hanno alzato la mano per intervenire è sempre stata data la parola. La possibilità di discutere su quegli articoli c'è stata. Il problema qual era? Eravamo fondamentalmente d'accordo su tutto. Quindi, oggi, per tentare di fare una piccola polemica, si cerca di sposare questa strada. La stessa cosa è accaduta alla Camera dei deputati, dove, anche lì a larghissima maggioranza,

incontro ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa, concedendo loro il giusto riconoscimento

dei doveri e dei sacrifici maggiori rispetto a quelli di altri tipi di funzioni e di altre categorie di dipendenti pubblici. È per tutti questi motivi che evidentemente annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

l'emergenza maltempo in questi giorni ha martoriato Valle d'Aosta e Piemonte, con danni infrastrutturali ai privati di grande portata. La macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente ed efficacemente. Ringrazio tutti i soccorritori e le istituzioni per il grandissimo lavoro fatto e che continuano a Ringrazio la popolazione valdostana e piemontese. I montanari sono per natura abituati a resistere di fronte a ogni difficoltà, stringendosi come comunità in cui tutti forniscono il proprio aiuto. Per questo la velocità con cui si sta rimettendo tutto in ordine nelle località colpite è impressionante. Chiedo al Governo di intervenire prontamente, ponendo le risorse necessarie per la ricostruzione e per far fronte ai danni patiti. Nel frattempo, aspettiamo tutti in Valle d'Aosta, pronta come sempre ad accogliere i turisti con calorosa ospitalità nel contesto incantevole delle nostre montagne. Signor Presidente, prendo la parola per lasciare, per il suo tramite, un promemoria al Ministro delle infrastrutture. In queste settimane sentiamo parlare molto di disagi, di ritardi sulle nostre linee ferroviarie, ma nessuno nessuno ha parlato di quello che è successo lo scorso fine settimana. Lo scorso fine settimana è successo qualcosa di assurdo. Un treno Intercity notte, il numero 1963, in partenza da Milano e diretto a Siracusa, è partito nella giornata di sabato 29 giugno

Nel treno c'erano all'incirca 150 persone che hanno raggiunto la destinazione di Siracusa con un ritardo incredibile, forse mai successo nella storia. Io capisco tutto, ma su questo tipo di situazione mi aspettavo almeno l'elaborazione di un pensiero da parte del Ministro delle infrastrutture, che invece non c'è stato. Già tempo fa, poche settimane fa, mi sono permessa di sollecitarlo per quel che riguarda l'assenza di una programmazione: una programmazione che avrebbe dovuto prevedere un numero maggiore di treni da e per la Sicilia, proprio in virtù della stagione estiva. però, non è avvenuto. Io mi aspettavo, Presidente, oltre chiaramente ad immaginarmi che la risposta del ministro Salvini sarebbe che con il Ponte si risolverà tutto *(Applausi)*, una parola da parte sua ultimi giorni, in queste ore, anche perché noi viviamo il presente e non il futuro. Diciamo che ogni volta che scendiamo da un treno ascoltiamo una voce registrata che ci ringrazia per aver scelto il servizio e ci invita a tornare sui treni Trenitalia. A mio avviso, con il ministro Salvini questo annuncio ha il sapore della beffa e, talvolta, della minaccia. *(Applausi)*.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 agosto. Nella seduta di domani, a partire dalle ore 17, sarà discusso il decreto-legge in materia di agricoltura e imprese di interesse strategico. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Nella giornata di giovedì 4 luglio, con inizio alle ore 10, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia alle quali seguirà la chiama. Ove concluso l'esame del decreto-legge, alle ore 15, si terrà il previsto *question time* con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e per le disabilità. La settimana dall'8 al 12 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Nella settimana dal 16 al 18 luglio saranno discussi i decreti-legge sulle liste di attesa in materia di ricostruzione e protezione civile. Per la giornata di martedì 16 luglio, eventuali votazioni si svolgeranno fino alle ore 17. Il calendario della settimana dal 23 al 25 luglio prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e la discussione dei seguenti decreti-legge: semplificazione edilizia e urbanistica; sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico; prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, ove presentato al Senato. Resta confermato il *question time* di giovedì 18 e 25 luglio, alle ore 15. Nella settimana da lunedì 29 luglio, alle ore 16, e fino a sabato 3 agosto, se necessario, saranno discussi gli eventuali argomenti non conclusi e i seguenti decreti-legge: materie prime critiche di interesse strategico; infrastrutture e investimenti strategici, processo penale e sport. Il calendario della settimana prevede altresì il disegno di legge sulla proroga del termine di adozione di testi unici in materia tributaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati. La settimana da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto, se necessario, prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi nelle settimane precedenti.